L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 marzo. Nella seduta di oggi sarà discusso il decreto-legge concernente la Presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati. Al termine sarà commemorata la figura di Franco Basaglia in occasione del centenario della nascita. Domani, alle ore 10, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR renderà comunicazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I tempi della discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi. Restano confermati gli altri argomenti già previsti per il calendario della settimana corrente e della prossima settimana, salvo il sindacato ispettivo del 21 marzo, che sarà sostituito dalla discussione di due mozioni, una proposta dai Gruppi di maggioranza e una dai Gruppi di opposizione. Il calendario dei lavori della settimana dal 26 al 28 marzo prevede la discussione dei seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali; dalla sede redigente, disegni di legge sulla promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia e sul contrasto del bracconaggio ittico; insindacabilità delle opinioni espresse da Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile presso il tribunale di Roma. Giovedì 28 marzo, alle ore 10, si terrà il sindacato ispettivo. D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori è convocata, per procedere alla sua costituzione, giovedì, 14 marzo, alle ore 13,30, presso la sede di Palazzo San Macuto. L'elenco dei componenti della Commissione sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione che ci apprestiamo a votare è cruciale per la buona riuscita del prossimo Vertice del G7, il *forum* che riunisce i *leader* dei 7 Paesi altamente industrializzati e di cui l'Italia ha assunto la Presidenza il 1o gennaio scorso. L'importanza di quest'evento è stata riassunta nelle poche semplici parole del Presidente del Consiglio pronunciate nel suo intervento di apertura di questa Presidenza: «Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e noi intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità». Come tutti ben sapranno, durante quest'anno sono previsti vari incontri ministeriali in diverse località italiane che toccheranno tutte le tematiche internazionali più scottanti (infrastrutture, trasporti, clima e ambiente, energia, finanza, finanza, ricerca, lavoro, agricoltura e salute). Il Vertice del G7, momento cruciale della Presidenza italiana, si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno e il provvedimento al nostro esame è finalizzato a farci trovare pronti per affrontare al meglio questo appuntamento.

con il compito di procedere alla realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali e manutentivi necessari allo svolgimento del G7 in generale e al Vertice dei Capi di Stato e di Governo in Puglia. Al fine di rendere il provvedimento più incisivo, è previsto che il commissario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti di cui all'articolo 1, La scelta di nominare un commissario è funzionale alla velocizzazione dell'affidamento per i lavori, che potrà avvenire attraverso procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara anche per gli appalti superiori alle soglie di rilevanza europea, solo per consentire la realizzazione degli interventi in modo tale da garantire l'operatività in vista del G7 e del Vertice. Ovviamente tale deroga deve essere supportata da una motivazione che, per singolo intervento, deve dare atto delle ragioni di necessità e di urgenza per le quali si deroga alla procedura ordinaria. fatto salvo il ricorso alla procedura di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. È infatti prevista al comma 2 la possibilità, per l'affidamento degli appalti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle reti stradali, che il commissario straordinario possa selezionare gli operatori anche nell'ambito degli accordi quadro stipulati dall'ANAS e ancora efficaci alla data dell'affidamento. Al comma 3 si prevede, sempre in un'ottica di velocizzazione dei tempi, la possibilità di anticipazione del contratto prima della stipulazione attraverso l'utilizzo degli accordi quadro conclusi e ancora efficaci da parte di ANAS per la selezione degli operatori e per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e della rete stradale. Per rispettare il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, si procederà secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 che, per la velocizzazione della procedura di verifica, prevede il ricorso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Poiché con questo provvedimento non viene lasciato nulla al caso, si prevede al comma 4 l'applicazione, nelle controversie che potrebbero sorgere sugli atti relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere di affidamento, dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Dunque, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo dell'urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi delle opere necessarie per lo svolgimento del G7 e del Vertice, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si deve tener conto della coerenza della misura cautelare adottata con l'urgenza della realizzazione dell'opera, ovvero degli interessi in gioco. Infine, per la realizzazione degli eventi di cui al comma 5, si dispone la deroga a ogni disposizione di legge, eccetto la legge penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le medesime previsioni di velocizzazione delle procedure sono poi estese all'affidamento dei lavori, servizi e forniture esperiti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli eventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la Presidenza italiana del G7. L'articolo 2 del provvedimento in discussione riguarda, come anticipato, la dotazione finanziaria per realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi, che ammonta a 18,050 milioni, incluso il compenso del commissario, che non può essere superiore a 50.000 euro, come previsto nel comma 1 dell'articolo 1.

È chiaro però che speriamo che questo decreto-legge, questo intervento economico di tipo organizzativo, serva anche a dimostrare un impegno nei confronti del G7. La nostra

stellare - per così dire - o splendida. Voglio per esempio ricordare che, quando nel maggio dell'anno scorso si è chiuso il G7 di Tokyo, nella cosiddetta foto di famiglia, nella fotografia che si fa alla conclusione di questi vertici, per l'Italia c'era l'ambasciatore Benedetti, perché la Presidente del Consiglio aveva deciso che aveva impegni più importanti in Italia. C'era stato il disastro dell'Emilia-Romagna la Presidente del Consiglio, probabilmente per poter cogliere una *photo opportunity,* ha indossato i suoi stivali di gomma, la sua giacca antipioggia e si è fatta fotografare in Emilia-Romagna. Purtroppo, però, il suo posto non era lì. Il posto del Governo era nel sostegno all'Emilia-Romagna che è arrivato con grande lentezza, quando è arrivato, nel senso che gli emiliano-romagnoli si sono dovuti rimboccare le maniche risolversi i problemi ben prima che arrivasse qualche fondo da parte del Governo. In compenso, però, la Presidente del Consiglio ha disertato la chiusura del G7 e ha dimostrato che probabilmente non era ancora nella condizione di cogliere l'importanza di essere presente in un consesso nel quale la creazione di rapporti e la possibilità di discutere grandi questioni internazionali, anche in una serie di bilaterali, richiedevano che in quella foto di famiglia ci fosse lei e non il nostro bravo ambasciatore Benedetti. Voglio però ricordare che, sempre durante quel G7, fu fonte di grande imbarazzo per la Presidenza del Consiglio, ma devo dire per tutto il Paese, il fatto che un altro dei membri del G7, il primo ministro canadese Trudeau, proprio nel bilaterale con Giorgia Meloni, in modo molto irrituale fece presente la preoccupazione del Canada - appunto un altro componente del G7 - circa la situazione dei diritti civili nella nostra Repubblica, in particolare dei diritti della comunità LGBT. un Primo Ministro di un grande Paese, un Paese importante come il Canada, in una situazione così formale, abbia tirato fuori una preoccupazione così seria e grave. La situazione deve essere

ben più accomodanti e accoglienti rispetto alle minoranze, è chiaro che si guarda all'Italia con una certa preoccupazione. Non può però sfuggire che il Canada è proprio uno di quei Paesi dove, per esempio, la gestazione per altri è molto severamente regolamentata, ma è lecita. Noi sappiamo che la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge, che proprio oggi - guardi i casi del destino, signora Presidente - abbiamo incardinato in Commissione giustizia al Senato, che prevede che i cittadini italiani che ricorrono alla gestazione per altri in Paesi dove è regolamentata e lecita, come il Canada, siano poi passibili di sanzioni penali una volta che tornino in Italia. Capisco bene l'imbarazzo di un Primo Ministro di un Paese sovrano come il Canada che si dà delle leggi e un altro Paese, come l'Italia, che dà in un certo senso delle patenti di inadeguatezza alla legislazione canadese, perché dice "guarda, caro Canada, se miei concittadini dovessero venire nel tuo Paese e rispettare le tue leggi sul tuo territorio,

in Commissione giustizia. Capisco bene lo sconcerto del primo ministro Trudeau e capisco anche che, quando un Paese come il nostro, di indiscussa civiltà giuridica, si trova a farsi tirare le orecchie in pieno G7 da un altro Paese, ciò sia fonte di imbarazzo. Speriamo che non accada a Borgo Egnazia e che il primo ministro Trudeau non tiri fuori qualcosa su qualche altro reato universale o sul grande numero di reati che questa

visto il viaggio della Presidente del Consiglio negli Stati Uniti, che credo sia servito anche a preparare il G7 in Puglia, e le prese di posizione condivisibili anche sulla guerra in Ucraina. Non sfugge a nessuno

divisa. Ricordo che sulle questioni legate all'Ucraina c'è almeno una forza politica della maggioranza che è molto tiepida, che è la stessa forza politica della maggioranza che, essendo pronta sempre a buttare la gente in prigione e a gettare via la chiave, ha scoperto il garantismo quando il povero Alexei Navalny è morto in Siberia; oltre il circolo polare artico,

se l'infrastruttura sarà pronta, molto bene. Mi sono permesso però in questo intervento in discussione generale di ricordare che l'infrastruttura, gli alberghi e le strade che dovranno condurre i *Leader* nel meraviglioso e ridente villaggio della Puglia saranno molto importanti, ma ancora più importante sarà il risultato del G7, come noi riusciremo a esprimere una *leadership;* una *leadership* che finora abbiamo espresso pochissimo sul piano internazionale. Basti guardare come è andata, per esempio, la gara per Expo 2030, dove soltanto 16 Paesi ci hanno votato, neanche tutti e 27 i Paesi dell'Unione europea. Avremmo tanti altri casi: l'Autorità antiriciclaggio, che è andata a Francoforte; il capo della Banca europea per gli investimenti, che non è stato Daniele Franco, nonostante la sua candidatura fosse di assoluto prestigio. Diciamo che sul piano della politica estera facciamo molta fatica. Speriamo che, mettendo a posto le strade, le infrastrutture e il cerimoniale, anche il resto segua e l'Italia colga l'occasione del G7 per fare una bella figura in tutto il mondo e non risulti un po' per così dire - l'anatra zoppa di quel gruppo che dovrebbe guidare e dare le proprie indicazioni e la propria ispirazione alla politica estera di tutto il mondo. **Saluto

con sette anni di anticipo che questo evento sarà ospitato dal nostro Paese e già da tempo sapevamo che doveva essere ospitato in Puglia.

a un commissario l'opportunità di fare quello che vuole. Stiamo, quindi, approvando una *deregulation* totale e nessun criterio, nemmeno quelli di sicurezza del lavoro, potrà essere controllato in tempi così brevi.

dove verrà ospitato il G7? Verranno concordate con la cittadinanza, con la Regione? Nulla di tutto ciò. Verranno rispettati i criteri antimafia, i criteri di sostenibilità, i criteri anticorruzione? Ci saranno gli appalti a cascata, quelli che avete voluto nel nuovo codice dei contratti pubblici? Avete revisionato

questo Paese e oggi andate a derogare il vostro codice degli appalti, che era proprio quello che voi avete approvato. *(Applausi)*. Quindi, negate sempre voi stessi. Vi rendete conto che siete la negazione di quello che fate? È una cosa assurda: siete bravissimi a negare quello che avete fatto pochi mesi fa. quindi presentato tanti emendamenti come al nostro solito, anche se il nostro lavoro spesso viene mortificato da questo Governo; in Commissione sono stati tutti respinti e, quando abbiamo chiesto rispetto a qualche emendamento, il Governo si è inventato - in questo siete bravissimi - una frase *passepartout*, valida per tutti gli emendamenti: "questo emendamento non è coerente con le finalità del decreto". Siete bravissimi: avete anche inventato una frase *passepartout* per giustificare il fatto che gli emendamenti e gli ordini del giorno nemmeno li avete letti. È per questo che parlavo di approssimazione.

per tanti emendamenti utili che davano garanzie di sostenibilità in termini di antimafia e di corruzione, emendamenti che sono stati bocciati. bocciati. Non vi rendete conto che questo modo di procedere è rischioso, perché anche i subappalti a cascata, in cui un'azienda vincitrice poi subappalta ad altra azienda all'infinito, comportano

è colpa di qualcun altro, perché il nuovo codice degli appalti l'avete approvato voi e prevede proprio questo meccanismo assurdo dell'appalto a cascata senza regole. quindi di un provvedimento pilatesco: cercate di dare sempre le responsabilità a un altro - in questo caso a un commissario - e invece il G7 poteva essere una grandissima opportunità. Se avessimo programmato prima questo intervento, avremmo potuto fare un dono alla mia Regione.

e, quindi, vi do il merito di aver scelto almeno un bel sito. Potevamo però donare a quel territorio delle opere che poi sarebbero servite anche dopo il G7.

quindi non ci saranno i tempi, perché la fretta è sempre sinonimo di cattiva qualità, di lavori fatti in maniera inadeguata.

Avevamo un nuovo codice degli appalti, ma anche in questo caso siete stati bravissimi ad aggirare le stesse regole che voi avete fatto. Complimenti e speriamo che almeno questo G7 possa non far sfigurare il nostro Paese agli occhi del mondo.

partendo dai suoi obiettivi, ovvero la necessità di assicurare l'organizzazione degli interventi infrastrutturali connessi alla Presidenza italiana. Il Vertice del G7 - come ricordato dal relatore - si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, tra pochi mesi, e tutti noi dobbiamo riconoscere l'importanza di questa occasione per il nostro Paese, peraltro in un momento di significative turbolenze geopolitiche. potremmo aprire - alcuni colleghi lo hanno fatto prima di me - un dibattito su come discutibili scelte politiche dell'attuale Governo abbiano portato a un isolamento crescente del nostro Paese nell'arena europea e internazionale, compromettendo questa grande opportunità. Noi, però, anche dall'opposizione, facciamo sempre responsabilmente il tifo per l'Italia e speriamo che il nostro Paese possa cambiare registro, affinché il G7 possa ancora rappresentare un'opportunità per rinnovare la nostra immagine globale e dare il nostro contributo per affrontare le grandi sfide che il mondo oggi si trova davanti. Questa maggioranza, però, non sembra così responsabile. Il G7 è nato nella prima metà degli anni Settanta del secolo scorso. Il primo Vertice dei Capi di Stato e di Governo, in formato ancora G6, risale al 1975; il formato attuale è nato nel 1976 con l'ingresso del Canada. Ogni anno - come ha ricordato il collega prima di me - a partire dal 1° gennaio uno degli Stati membri assume a rotazione la guida del gruppo. Sono passati quindi quasi cinquant'anni e questa è la settima volta che l'Italia ne assume la Presidenza. Vista l'urgenza del decreto-legge in esame, dobbiamo però constatare che non vi è bastato il preavviso di cinquant'anni per prepararvi. Decisamente dovete cambiare *slogan*: non potete più usare quello di essere pronti. Ma non solo: queste deroghe per il G7 non fanno che confermare il *bluff* di un Governo che solo pochi mesi fa presentava con grande enfasi una riforma del codice degli appalti come chiave per un futuro di efficienza e di crescita. La realtà, tuttavia, dimostra che tali promesse erano illusorie e che le scelte operative attuali sono lontane dagli enunciati principi di semplicità, velocità e riduzione della burocrazia. Avete introdotto gli appalti a cascata e peggiorato le condizioni di sicurezza per i lavoratori, con passi indietro significativi sulla parità di genere e sull'occupazione femminile, sui cittadini e sul mondo dell'impresa sano, che ha tutto l'interesse a confrontarsi in un sistema dove prevale il rispetto delle regole. Eppure, il vostro nuovo codice degli appalti non è mai in grado di far fronte a nessun impegno. Oggi, la decisione contenuta in questo decreto di derogare per l'ennesima volta al codice degli appalti, semplificando persino i controlli antimafia, rappresenta un passo indietro significativo per la trasparenza e l'integrità del nostro sistema. Questa scelta conferma quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero un approccio del Governo ai lavori pubblici inefficace e contraddittorio. Per questo, signora Presidente, pur sostenendo la necessità di organizzare al meglio il G7 nel nostro splendido Paese e di utilizzare questa opportunità per promuovere l'Italia sulla scena internazionale, dobbiamo esprimere la nostra contrarietà al provvedimento in discussione. Le modalità scelte per la sua attuazione, in particolare la deroga al codice degli appalti con semplificazione dei controlli antimafia, rappresentano un chiaro passo falso. Queste decisioni, insieme alla totale chiusura a proposte emendative costruttive, possono minare gli sforzi di ristabilire la credibilità dell'Italia agli occhi del mondo. Il nostro auspicio è che l'intero *iter* procedurale si realizzi in totale assenza di anomalie o passaggi opachi perché, nella malaugurata ipotesi che, al contrario, intervengano problemi, il danno di immagine sarebbe irreparabile. In definitiva, signora Presidente, mentre il G7 potrebbe essere un faro di speranza per il nostro Paese, questo decreto rischia di spegnere quella luce prima ancora che possa brillare. È il momento di riconoscere che l'integrità, la legalità, la trasparenza e la responsabilità sono non opzionali, ma la vera chiave per un futuro in cui l'Italia possa orgogliosamente mostrare la sua bellezza, forza e ingegno sulla scena mondiale.

Signora Presidente, fondamentalmente, quello che viene sacrificato con questo metodo di lavoro basato sull'urgenza è anche l'impatto ambientale degli interventi. Nel mio emendamento 1.29 sottolineo sottolineo l'importanza di un monitoraggio e di una valutazione delle impronte di carbonio idrica ed ecologica. Quindi, chiedo che in fase iniziale, ma soprattutto in fase conclusiva di questo evento, vengano vengano pubblicati questi dati, in modo da poter monitorare quale sia l'impatto, quali siano le criticità che eventualmente emergono, in modo da poter lavorare successivamente anche in pianificazione.

lavori con maggior rapidità per rendere più confortevole e agibile il G7 in Italia. Nonostante la semplicità del provvedimento,

i propri indirizzi e le proprie sensibilità e attitudini rispetto a un provvedimento di questo genere. Penso però che la cosa più importante sia il fatto di poter andare incontro alla possibilità di creare una vera cartolina di quella che è l'Italia attraverso attraverso il miglioramento delle infrastrutture, per poter rendere il più agevole e confortevole possibile a tutti quanti i partecipanti del G7 il soggiorno in essa, mostrandola agli occhi del mondo nel miglior modo possibile. Abbiamo una cornice naturale spettacolare, che è quella della Puglia, che naturalmente rende molto più facile questo tipo di lavoro. L'aspetto più importante però è quello politico, la centralità che ha riassunto l'Italia nell'ultimo periodo da un punto di vista

se, a dir la verità, c'era tutto il tempo per evitare un decreto d'urgenza con misure straordinarie, posto che l'Italia era a conoscenza da tempo avete avuto un anno e mezzo per poterlo preparare. Per non dare però alibi alla destra del Governo del Paese di dire che non si vuole bene alla Nazione; che vogliamo farle fare brutta figura; che non siamo collaborativi

che ci sia un'esplicazione su cosa il nostro Paese andrà a dire in tutti i s*ummit* che avete previsto e poi in quello finale, ovviamente, in Puglia. Lo dico perché mi ha molto colpito, ad esempio, che uno dei primi momenti di riflessione del G7 sarà sull'intelligenza artificiale. Mi ha colpita questo elemento perché la scorsa settimana, in audizione in 8a Commissione, è venuto l'amministratore delegato della TIM a esplicitare la

e casualmente - questa è la grande sorpresa - il Governo non ha azionato la *golden power*: possibilità che era data da un DPCM firmato Gentiloni e

aveva individuato la rete telefonica come prioritaria per lo sviluppo del nostro Paese e il Governo sovranista guidato dalla Meloni non aziona la *golden power* e permette di vendere la rete agli americani.

Inoltre, i soldi della vendita della rete non serviranno neanche a ripianare i debiti di TIM, e nel contempo abbiamo perso una grande infrastruttura. alla mia domanda. Nella prima riunione nella quale si parlerà di intelligenza artificiale, a parte la solita - giusta - lamentazione europea, secondo cui l'Europa è messa a lato perché è una partita che purtroppo si giocano soltanto gli Stati Uniti e l'Asia (in particolare la Cina),

che la *golden power* venisse applicata e la rete venisse considerata un'infrastruttura strategica. Oggi approviamo la cornice

temo che in quell'occasione il nostro voto non sarà favorevole, perché è bastato questo esempio, relativo alla rete, per dimostrare come a parole i sovranisti siano bravissimi a far campagna elettorale ma, una volta andati al Governo, svendano il Paese peggio degli altri Governi.

si avvale per l'ennesima volta della logica emergenziale utilizzata impropriamente dal Governo Meloni anche in questa occasione, nella quale è impegnato a confrontarsi su temi cruciali con i *leader* dei Paesi che si riuniranno in Puglia dal 13 al 15 giugno prossimo. Nel provvedimento si legge che il regime derogatorio con cui si intendono gestire i lavori connessi all'organizzazione di questo incontro e delle successive riunioni ministeriali che si terranno in varie località italiane sino alla fine dell'anno è giustificato dalle strette tempistiche di realizzazione; tempistiche indubbiamente strette oggi, ma solo perché si è deciso di non fare niente ieri. La Presidenza del G7 ruota, infatti, di anno in anno; quella assunta dall'Italia non è capitata improvvisamente tra capo e collo, ma è ben nota già a partire dall'anno scorso. Ricordo alle colleghe e ai colleghi della maggioranza che l'annuncio del luogo che ospiterà il Vertice è stato dato dalla stessa *premier* Meloni già dallo scorso maggio. Arrivare a marzo di quest'anno, a soli due mesi dall'evento di giugno, per discutere gli interventi infrastrutturali e decretare d'urgenza per il G7 è semplicemente scandaloso: è un segnale evidente che anche in questa occasione l'Esecutivo manca di una puntuale e competente programmazione dei lavori, operando in un'ottica del fare tutto all'ultimo momento, tanto siamo nel Paese *open* alle deroghe nel quale le mille eccezioni non confermano la regola, ma vanno bensì ad annacquarla, ad annegarla e a negarla. Così, anche il decreto-legge in esame non rappresenta uno splendido e memorabile esercizio di buona politica da parte del Governo Meloni, che tutto fa tranne che orientarsi verso una modalità operativa più consona alle sfide da affrontare oggi e per il futuro del Paese; modalità che richiede sicuramente una transizione di mentalità, data anche dall'agire per tempo e non fuori tempo. Ciò vale per la transizione ecologica, per quella energetica, per il contrasto al dissesto idrogeologico, per la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, eccetera. Agire per tempo è ancora possibile e, quindi, invito il Governo a un deciso cambio di rotta. Tornando al provvedimento in esame, con lo stanziamento di 18 milioni di euro, il decreto-legge affida a un commissario straordinario il compito di procedere all'urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi relativi al G7; caso l'ennesimo commissario straordinario - e io pago, come diceva già Totò - i cui costi graveranno sulle casse dello Stato e quindi sui cittadini. Abbiamo ormai perso il conto delle nomine di commissari da inizio legislatura, tanto che ci si chiede come sia possibile districarsi in questa giungla amministrativa, come viene monitorato il loro lavoro e se veramente sono funzionali al compito loro ascritto. È evidente che questo Governo, oltre che amare le deroghe, fa anche uso e abuso di personalità tuttofare incaricate di guidare in fretta e furia procedimenti altamente delicati come quelli relativi all'affidamento degli appalti, nominati per svariate emergenze - che emergenze non sono - dall'inizio della legislatura.

o alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, in deroga rispetto alle soglie di rilevanza previste dal diritto europeo, o all'affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici; tutto ciò esigendo che l'esecuzione dei contratti avvenga prima della stipula e applicando, per quanto attiene alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia, la norma semplificatoria adottata nel contesto emergenziale della pandemia, che prevede il solo rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria a garanzia delle verifiche antimafia e del rispetto dei protocolli di legalità nell'esecuzione dei contratti. Peccato che la pandemia sia finita, e non invece questa politica e questa pratica emergenziale trascinate ormai anche per la gestione di un evento internazionale. Queste sono disposizioni derogatorie insostenibili e incomprensibili, che aprono di fatto un varco alle infiltrazioni criminali nella scelta delle società appaltanti; decisione ancora più grave se si pensa che tale deroga è estesa a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, in modo totalmente indefinito anche nella fase di affidamento e di esecuzione dei lavori. Ricordo, a questo proposito, che persino il Comitato per la legislazione della Camera si è espresso in maniera critica su questo punto, segnalando l'opportunità e l'onere del legislatore di circoscrivere meglio i limiti di tale deroga. Insomma, un "libera tutti" francamente non comprensibile che, invece di rafforzare il rispetto dei principi di affidabilità, trasparenza e sostenibilità, anche ambientale, dei lavori, definiti normalmente dal nostro codice degli appalti e dalla normativa europea, punta unicamente al risultato di facciata, bypassando la verifica del rispetto di ogni presidio di legalità. Da qui il nostro lavoro emendativo, con cui abbiamo cercato di ammorbidire l'approccio proposto, naturalmente non accettato. È imbarazzante constatare che, a fronte dei temi che verranno trattati nell'ambito dei lavori del G7, manchi in questo provvedimento una visione che contempli il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici dell'esecuzione delle opere. Così come è imbarazzante che la Presidenza italiana ponga all'ordine del giorno argomenti come il cambiamento climatico e il nesso clima-energia, rispetto ai quali il G7 ha la responsabilità e il dovere di individuare, insieme ai suoi *partner* globali, soluzioni innovative, per poi trascurarli totalmente nella realizzazione delle strutture che ospiteranno i dibattiti, rischiando di fare una vera figuraccia a livello internazionale. un comportamento incoerente e inconsulto, che non dobbiamo né possiamo accettare. Anche per questo abbiamo proposto degli emendamenti che stabiliscono il rispetto dei criteri minimi ambientali inseriti nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e individuati dal piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, la cui efficacia è garantita dallo stesso codice degli appalti. Inoltre, al fine di orientare gli interventi infrastrutturali del G7 al rispetto dei criteri ambientali, abbiamo proposto di utilizzare l'indicatore del c*arbon footprint*, ossia del calcolo delle emissioni dirette e indirette delle opere, come criterio di scelta nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, sull'esempio di quanto fatto dalla Presidenza tedesca che, nell'anno 2022, ha organizzato il G7 a Schloss Elmau in Baviera. Adottando un programma organizzativo improntato alla sostenibilità e all'abbattimento delle emissioni connesse allo svolgimento degli eventi, la Presidenza tedesca ha garantito il rispetto di specifici *standard* ambientali nell'organizzazione degli incontri, dando un importante segnale di coerenza anche rispetto alle decisioni politiche adottate in materia di clima e ambiente in quella sede. È un segnale che il Governo Meloni non vuole dare. Sebbene l'Italia sia perfettamente in grado di garantire gli stessi *standard* in questa importantissima occasione di dialogo e confronto con i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi tra i più avanzati e industrializzati al mondo, è evidente che l'Esecutivo Meloni non intenda organizzare il G7 nel rispetto di tali criteri minimi ambientali. Peccato che non abbia intenzione di dimostrare che anche le infrastrutture che ospiteranno le delegazioni possono essere perfettamente in grado di rispettare gli stessi criteri di sostenibilità ambientale che i Paesi del G7 si impegneranno a perseguire nella loro attività politica e legislativa. Un'altra occasione sprecata, un altro evento di facciata. Perciò questo provvedimento va in una direzione totalmente opposta rispetto a quella da noi proposta e, quindi, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra dichiariamo il nostro voto contrario.

- polemiche sulle procedure d'urgenza che oggi si devono attuare per poter mettere in sicurezza i luoghi sensibili, perché ci saranno le sette potenze mondiali e i sette *leader* sul nostro territorio in Italia

ad esempio con l'ANAS. Non vedo nessuno scandalo e non capisco perché scandalizzarci davanti a procedure d'urgenza che forse possono essere utili nel nostro Paese per fare sempre più e migliori opere pubbliche.

in un momento particolare per il nostro Paese, con tutto quello che sta succedendo alle porte dell'Italia, nell'area del Mediterraneo e dei Balcani, e con il conflitto russo-ucraino alle porte dell'Europa. Quindi, è un momento sicuramente delicato. Rifacendomi

Si tratta di un territorio che - come dicevo - si affaccia e fa da ponte verso i Balcani, verso l'Oriente e soprattutto verso il Nord dell'Africa, che in questo momento svolge anche un ruolo

20 milioni di euro per l'allargamento delle aree esterne, il potenziamento delle *control room* e della *security*, i varchi o le aree esterne dei *terminal*, l'implementazione delle reti.

per l'Italia tutta. Come dicevo, la Puglia che si affaccia sui Balcani può svolgere un ruolo internazionale molto importante. È la Puglia del turismo e dell'agroalimentare che conosciamo, e non solo. Ecco perché il G7 è un'opportunità

della nostra Puglia; un'occasione storica per tutta la Puglia, per il Sud, per mostrare al mondo intero le capacità e le potenzialità enormi del territorio. È proprio a questo che mira il decreto-legge al nostro esame, perché il provvedimento che oggi approviamo disciplina la nomina e i poteri del commissario straordinario che realizzare gli interventi infrastrutturali e soprattutto manutentivi. La scelta di affidare tali interventi a un commissario è funzionale alla celerità degli interventi che devono essere messi in campo e quindi è un banco di prova importante. Ci saranno delle gare veloci, che utilizzeranno già

e stradali, ci sarà la collaborazione di ANAS. Per la realizzazione di questi interventi si procederà in deroga alle disposizioni di legge:

riguarda le ricadute infrastrutturali dei lavori necessari a supportare l'evento, che sono stati concertati con le realtà locali. Quindi, oltre al supporto tecnico-amministrativo

primo passaggio alla Camera. Il Gruppo Forza Italia ha lavorato alacremente proprio per apportare dei contributi, come sempre facciamo su tutti i provvedimenti, e i contributi sono volti anche a tenere conto delle realtà del territorio pugliese e della possibilità di lavorare con il nostro territorio. Saranno a disposizione anche le autorità portuali del territorio della nostra Puglia, che daranno un contributo, così come tutte le autorità oggi presenti in Puglia. Si tratta di un provvedimento al quale abbiamo lavorato tutti quanti con grande attenzione. Lo abbiamo fatto anche migliorandolo, come Gruppo Forza Italia. Io lo faccio anche - consentitemi - con grande partecipazione emotiva, perché è un evento importante che dà lustro sicuramente a tutta l'Italia, sicuramente al nostro Paese, che sarà centrale in quei giorni a livello mondiale e poi - come dicevo - anche e soprattutto per la mia amata Puglia. È per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

nel preannunciare il voto sfavorevole del MoVimento 5 Stelle, vorrei osservare al collega che mi ha preceduto che non è nostra intenzione sminuire l'evento del G7 in sé. sé. La nostra critica è rivolta alle modalità e alle tempistiche con cui questa maggioranza e questo Governo stanno gestendo un evento di cotanto rilievo e importanza internazionale. Mi piace citare le parole della presidente Meloni: abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e vogliamo onorare questo impegno al massimo delle nostre possibilità. Siamo Siamo a metà marzo: l'evento si svolgerà i primi di giugno e il massimo delle nostre possibilità è avere due mesi per organizzare un evento così importante,

Si lavora in emergenza. Un detto popolare recita che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi e di solito c'è da fidarsi dei detti popolari. Si ricorre quindi a un commissario straordinario straordinario e alle deroghe. Chiaramente, per poter lavorare in velocità, occorre eliminare tutti gli ostacoli che potrebbero frapporsi tra noi e il raggiungimento di questi obiettivi che, tra l'altro, ancora non si capisce bene quali siano. Saltano allora i bandi di gara,

nell'ottica della velocizzazione. Vietato fare qualsiasi proposta per non appesantire, non infastidite il manovratore. Solo che - ahimè - senza le garanzie e derogando a tutte le tutele, rischiamo, come al solito, di creare danni anziché benefici. Sono state chiaramente respinte anche le misure contenute negli ordini del giorno: l'auspicio che venissero presi in considerazione i criteri minimi ambientali, la *carbon neutrality*, la valutazione di quello che resterà sul territorio in conseguenza di questi interventi (per esempio in termini di impronta di carbonio, idrica o ecologica). Conosciamo i tempi in cui viviamo e sappiamo che bisogna prestare attenzione a tutte le modifiche che vengono apportate al territorio nell'ottica della prevenzione del dissesto idrogeologico e di tutto quello che tali interventi possono comportare. Poteva essere questa un'occasione, una vetrina

di questi obiettivi. Per il momento però non si sa nulla. Tutti i nostri emendamenti, le nostre osservazioni e i nostri contributi non sono stati presi in considerazione. Non appesantire, avanti così e buona fortuna all'Italia. Mi auguro solo che in questa occasione internazionale in cui si svolgerà questa vetrina non si venga a ripetere l'increscioso episodio di cui sono stati protagonisti la nostra Presidente del Consiglio e il presidente Biden, in occasione di una visita alla Casa Bianca della presidente Meloni. Mi riferisco a quel bacetto sul testolino del nostro Presidente del Consiglio, quel bacetto paternalistico, ma soprattutto alla reazione del nostro Presidente del Consiglio, che ha abbassato lo sguardo e ha fatto un sorrisino imbarazzato. Da madre, da donna e da italiana, mi permetto di osservare che una donna in quella situazione avrebbe ben potuto fare un passo indietro, recuperare le distanze fisiche e mediatiche, allungare il braccio con una mano aperta in cerca di una stretta di mano di una vigorosa stretta di mano. Quel gesto e quella reazione sono infatti sintomo di una fragilità estrema. Il nostro Presidente del Consiglio dovrebbe sapere che, per guadagnarsi i virtuali attributi, non basta declinarsi al maschile: bisogna anche comportarsi in modo da ottenere il rispetto e garantire agli italiani la dignità. *(Applausi)*. Mi auguro quindi che anche l'aspetto infrastrutturale, mediatico e mentale

Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per il Gruppo Lega-Salvini Premier e lo faccio

un momento storico in cui l'Italia si trova ad ospitare i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, Uniti, in un momento particolarmente delicato della storia globale. Si parlerà delle guerre in corso, ma anche di questioni migratorie e sarà all'attenzione dei lavori del G7 anche il tema dell'intelligenza artificiale. Proprio il prossimo 15 marzo saranno a Trento per la riunione ministeriale su industria e tecnologia i Ministri dei sette Paesi più industrializzati del mondo, fra i quali - è bene ricordarlo - dal 1997 al 2013 c'è stata anche la Federazione Russa, a titolo semplicemente diplomatico e in

nella maniera più educata, elegante e, in questo caso, più istituzionale possibile. Mi genera qualche meraviglia, tutta l'attenzione verso la nomina di un commissario e verso la necessità di portare a termine alcune semplici opere. È giusto ricordarne la natura, perché qui sembra che stiamo parlando di una rivoluzione copernicana, stiamo parlando della messa in sicurezza di 147 chilometri complessivi su varie arterie suddivise fra strade comunali, provinciali e statali; stiamo parlando della realizzazione di elisuperfici che completano e saturano le proposte infrastrutturali per accogliere i nostri ospiti. Nessuno ha parlato, invece, delle grandi attività che dovranno svolgere anche le amministrazioni locali, perché

di questa struttura che non ha un'organizzazione permanente e che naturalmente vede la Nazione che presiede questo consesso ospitare i lavori e i Capi di Stato e di Governo. Fra i vari appuntamenti ce n'è uno in particolare che genera in me molta emozione e sono lieto che si possano spendere anche i pochi soldi velocemente con un commissario. Uno degli eventi più importanti - mi sia permesso

una serie di giornate dedicate alla disabilità nella sede del G7 - vedrà per la prima volta i sette grandi sedersi a un tavolo nella Regione Umbria. Mi sembra peraltro che i lavori partiranno proprio dalla città di Assisi, portando anche grande rispetto per quella figura che tutti noi, nei nostri cuori e nelle nostre parrocchie, siamo spesso vocati a ricordare con una preghiera. Proprio nella città di san Francesco si inizierà a parlare di strategie e di impegni per contrastare le discriminazioni e garantire alle persone disabili pieno diritto alla partecipazione civile, sociale e politica. quindi il ministro Locatelli e tutti gli altri Ministri che si faranno parte attiva per organizzare degli eventi similari. Questo in particolare, però, è molto più importante perché indica che gli altri *partner* hanno voluto accettare, nell'ambito dei rapporti relazionali, anche una particolare attenzione verso quel tema tanto caro a molte famiglie, a molte associazioni, ovvero quello delle disabilità che i Paesi più sviluppati, più industrializzati, non possono certo trascurare. intervento rigettando ai destinatari quelle terminologie che ho sentito utilizzare: svendita del Paese, gestione scorretta degli appalti, piani piani che sarebbero stati velocemente raffazzonati per tamponare esigenze che potevano essere tranquillamente gestite in via ordinaria. Beh, non è così, e lo ripeto:

decoro e l'immagine del nostro Paese e a dimostrare che, quando qualcuno viene a casa nostra, siamo degnamente in grado di ospitarlo facendo trovare un ambiente accogliente, un caminetto acceso, un piatto di minestra sul tavolo e magari un po' di pulito intorno. Si tratta solo di questo: si chiamano educazione e cultura dell'accoglienza. Visto che di accoglienza ci parlano sempre molto i nostri amici della sinistra, stavolta diamo dimostrazione di essere veramente molto accoglienti, naturalmente con chi bussa alle nostre porte in maniera altrettanto educata. ancora una volta il Parlamento viene pressoché escluso dalla conversione in legge di un decreto-legge. Rispetto agli altri, questa volta il provvedimento riguarda gli interventi infrastrutturali per la settima Presidenza italiana del G7 che cade in un periodo complesso, di gravi tensioni internazionali e di grandi sfide per il Paese e per l'Europa: dall'energia alla transizione verde, dall'intelligenza artificiale all'autonomia strategica dell'industria europea. L'Italia si prepara a ospitare gli eventi del G7, anzitutto il Vertice di Fasano del prossimo giugno. Tuttavia, al Parlamento non è stato concesso né il tempo né il modo di collaborare attivamente, di partecipare alla predisposizione delle norme per le relative misure infrastrutturali.

che di fatto può rallentare ma non limitare la procedura negoziata in relazione all'affidamento degli appalti per gli interventi connessi al G7. Insomma, ancora una volta c'è un errore marchiano del Governo, anzitutto di metodo: in pratica, l'Esecutivo pone stretti confini all'azione di controllo proposta del Parlamento, e ciò in un ambito di estremo rilievo, come se nulla avessero insegnato gli sprechi enormi per il G7 del 2009. Guarda caso - forse è solo un caso, al Governo allora c'era sempre il centrodestra e a distanza di quindici anni rimane identico a se stesso, sia per i rapporti con il Parlamento sia per la gestione degli eventi che ci espongono e ci impegnano a livello internazionale. Stavolta, però, la Presidenza italiana del G7 è un appuntamento ancora più importante, dati i conflitti internazionali, i cambiamenti, gli equilibri politici ed economici nello scenario internazionale. L'Italia ha, dunque, un'opportunità unica per riaffermarsi sul palcoscenico internazionale che però il Governo sottovaluta, anche alla luce delle criticità amministrative e finanziarie contenute in questo decreto-legge relativo alla gestione dei preparativi del G7. Desta forte preoccupazione la scelta di affidare la gestione degli interventi infrastrutturali a un commissario straordinario, centralizzando ancora le decisioni. Questa scelta, che peraltro è l'ennesima di una lunga serie, esclude concretamente dai processi decisionali decisionali il Parlamento, ma anche e soprattutto le amministrazioni locali e gli enti territoriali, che invece hanno conoscenza diretta delle esigenze e delle priorità del territorio. Ogni territorio deve avere voce in capitolo nelle decisioni che lo riguardano direttamente. Ma il centrodestra non lo ammette: non vuole e non è disposto ad accettarlo, come abbiamo visto sulle questioni molto delicate, come per il tema dell'energia. Inoltre, stando a questo decreto, la procedura negoziata, cioè senza bandi cioè senza bandi per l'affidamento degli appalti, solleva seri dubbi sulla trasparenza e la competitività del processo, aumentando il rischio di favoritismi e di inefficienze. Ritengo particolarmente grave e preoccupante - come è stato sollevato dal collega Basso in discussione generale - la deroga alla normativa antimafia che potrebbe compromettere l'integrità delle procedure di assegnazione e realizzazione degli interventi.

Anche le questioni finanziarie non sono irrilevanti. L'importo stanziato di 18 milioni di euro solleva interrogativi sulla sua adeguata distribuzione e sulla reale necessità di alcuni investimenti, come le due elisuperfici.

è il vero aspetto critico. L'opposizione - in particolare noi del Partito Democratico - aveva fatto delle proposte emendative, specialmente in merito alle *white list*, per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle imprese coinvolte. Questa chiusura al dialogo è ancora una volta emblematica e conferma che il Governo vuole agire da solo, sempre da solo, tenendo a distanza il Parlamento e i territori. Di fronte alle criticità di questo decreto avevamo proposto degli emendamenti volti ad aumentare le risorse disponibili, a valorizzare il patrimonio pubblico, a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a controllare meglio i fornitori scelti, a potenziare le infrastrutture utili della Puglia. Se non bastasse, però, abbiamo presentato ordini del giorno per garantire trasparenza, tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche a esclusivo beneficio della collettività.

pubbliche. Però, anche se noi abbiamo fatto tutto questo, poco si realizza, quando dall'altra parte manca l'interlocutore che anche in politica estera mostra superficialità e ambiguità smisurate. Il Governo avrebbe dovuto riconsiderare il suo approccio rispetto all'organizzazione della Presidenza italiana del G7, promuovendo ampie trasparenze e il coinvolgimento degli amministratori locali. Si dovrebbe lavorare insieme per l'Italia, affinché sia *leader* in Europa e nel mondo. Il Governo, però, è sordo su tutto. Insomma, si tratti di G7, si tratti di qualunque lavoro pubblico in Italia, per voi non cambia, come per il codice degli appalti, che prima ostinatamente avete cercato di difendere e poi, con un colpo di penna, in questo decreto avete cancellato. La verità la storia degli ultimi due anni, quasi due anni di Governo, dimostrano che siete totalmente allergici alla condivisione e alla trasparenza. Anche per questo, noi votiamo no Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, è con grande gioia che mi accingo a fare la mia dichiarazione di voto su questo provvedimento che per noi pugliesi - e mi rivolgo al presidente Boccia, anche lui pugliese - significa tante cose insieme: significa potenziamento della rete stradale e dei sistemi di trasporto, nuove infrastrutture informatiche, opere di sicurezza, promozione turistica, sviluppo delle imprese locali, valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico, visibilità internazionale. In Puglia, in quasi vent'anni di Governi di Governi regionali guidati dal centrosinistra, non si sono mai visti così tanti interventi tutti insieme, opere che avranno un impatto economico diretto e indiretto a lungo termine: un'eredità che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ecco perché, presidente Boccia, da pugliese che vive nella sua Puglia, dove sono le mie radici, la mia famiglia, la mia attività politica, non posso che essere fiero che il G7 porti i grandi del mondo proprio nella mia Regione. Un'occasione migliore non poteva capitare e di questo ringrazio il presidente Meloni, il rappresentante del Governo, il relatore Gianni Rosa, esempio di laboriosità oggettiva. Quell'immagine stilizzata di un ulivo secolare, scelto quale *logo* della Presidenza italiana del G7, farà il giro del mondo. È l'ulivo pugliese che interpreta il nostro spirito: abbiamo radici profonde, ancorate nella tradizione, e fronde rigogliose proiettate nel futuro verso le sfide globali; lo stesso ulivo

La scelta strategica della Puglia denota, dunque, quella straordinaria e quotidiana attenzione che questo Governo ha per il Mezzogiorno. Tante bugie Tante bugie sono state dette in questi mesi. L'opposizione strumentalizza qualsiasi provvedimento, qualsiasi iniziativa. Perfino un *post* o un video sui *social* diventa oggetto di critica o di interrogazioni parlamentari. Per non parlare di quello che si è detto sull'autonomia differenziata che, visti gli strafalcioni scritti e detti da gran parte delle opposizioni, moltissimi hanno commentato senza finire di leggere neanche l'articolo 1. si possa affermare con granitica certezza che il Governo Meloni stia dando seguito e concretezza alle idee per cui i cittadini ci hanno votato, rendendoci il primo partito in Italia. Per questo ringrazio e saluto i colleghi Sigismondi e Liris, che sono stati interpreti della vittoria di qualche ora fa in Abruzzo. Vorrei ricordare a questa Assemblea che proprio nel giorno in cui il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia a questo Parlamento, ha ribadito, tra le altre cose, l'impegno determinato del Governo a sostenere le Regioni del Sud, un Sud visto non più come un problema,

Le infrastrutture sono un punto focale del decreto: è infatti previsto un piano strutturale in grado non solo di soddisfare le esigenze immediate del *summit*, ma anche di lasciare un'eredità positiva e senza precedenti nel nostro territorio. Questo provvedimento si iscrive in un quadro di preparativi che va oltre l'aspetto infrastrutturale, contemplando anche la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo, sottolineando il suo ruolo di Paese ospitante a livello diplomatico e culturale. è pronta a dimostrare ancora una volta di essere il crocevia ideale e naturale per un dialogo internazionale e a offrire l'accoglienza e l'eccellenza tutte italiane. non può che ritenersi una sfida, un'opportunità, un'occasione che dovrebbe riguardare tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. È un impegno e, ritengo, anche una responsabilità di tutti che riguarda il bene della nostra Nazione, il mondo dell'economia, del lavoro, del sindacato, delle imprese, delle associazioni di categoria, del terzo settore, del sociale. Chiunque si occupi della cosa pubblica dovrebbe tifare per il Governo; dovrebbe tifare per una riuscita impeccabile del *meeting* mondiale; dovrebbe tifare per l'Italia. Come quando gioca la nazionale di calcio, non possiamo e non dobbiamo essere divisi su questo, perché puntiamo lo dovremmo fare tutti - allo stesso obiettivo. L'Italia finalmente torna ad essere protagonista. È un'occasione per rimettere in primo piano la strategicità del mar Mediterraneo. Questo Governo ha dovuto fare i conti con un contesto internazionale problematico e sfidante, con una complessa situazione economica, con margini di bilancio limitati e con l'esigenza di garantire la coerenza dico «coerenza», parola quest'ultima non sempre cara a tutti - che ha confermato una solida e centrale collocazione internazionale del nostro Paese. L'Italia torna a parlare e soprattutto a far sentire la propria voce. Torna al centro dell'Unione europea su moltissimi temi, come la gestione dei flussi migratori, puntando sul tema del rafforzamento delle frontiere esterne e sulla collaborazione con i Paesi terzi. Gli accordi con la Tunisia e l'Albania, seppur diversi per contenuti e finalità, sono la testimonianza di questo approccio. Il Piano Mattei - ringrazio il senatore Rosa Rosa - è un ambizioso progetto, è la fotografia nitida della speciale attenzione che si è voluta dedicare al tema dei rapporti con l'Africa, un continente che noi consideriamo importante per la straordinaria potenzialità in termini di risorse energetiche e di materie prime, ma anche come *partner* con cui cooperare. Finalmente l'Italia torna protagonista in Europa e nel mondo. La Puglia sarà all'altezza di questa sfida, con l'invito a tutte le forze politiche e ai rappresentanti istituzionali del territorio di fare squadra ripeto: fare squadra - mettendo da parte steccati ideologici e preconcetti, per dimostrare che la Regione Puglia e la nostra Italia hanno le capacità e le risorse per guidare il G7 e affrontare le sfide che il mondo ci impone. Con questo provvedimento il Governo Meloni ha dato alla Puglia un'ala di riserva. Parafrasando una celebre preghiera di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, con questa seconda ala la nostra Regione è pronta a spiccare il volo con orgoglio e determinazione. Per tutti questi motivi, con gioia e soddisfazione, esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è convertito

onorevoli colleghi, come spesso mi accade quando parlo di qualcuno che a livello terrestre non c'è più, ma che è in noi tutti, nelle nostre anime e nei nostri comportamenti, un po' parte del mio carattere, esprimo pensieri che condivido e - come disse Woody Allen - pensieri che non condivido: la tristezza la malinconia di non avere più un maestro di tal fatta; la gioia o, meglio, la serenità di vedere affermate in maniera concreta le sue, le le nostre battaglie per far diventare la persona con sofferenza mentale una persona al centro dei nostri interessi e non l'oggetto da sorvegliare e punire (soprattutto le donne) nelle fosse dei serpenti di allora, nei manicomi,

molto ripida, soprattutto nella nostra mentalità che tende a costruire ancora steccati, sbarre e letti di contenzione anzitutto psicologici.

con professionalità ci ha condotto tutti, infermieri psichiatrici, medici, familiari di persone con sofferenza mentale, a fare una battaglia di civiltà: chiudere gli ospedali psichiatrici.

Franco Basaglia è stato fermamente dolce. Io ci ho persino litigato affermando la mia voglia di dedicarmi...

Il resto lo stiamo facendo adesso, celebrando in questa Aula sicuramente un grande tecnico, un politico, che non si è mai fatto affascinare dai partiti, ma che ha vinto assieme a noi, con dolcezza, una fase fondamentale, quella della chiusura dei manicomi. Il resto sta a noi: migliorare le leggi di salute mentale,

Signor Presidente, è con una certa emozione che ricordo la figura di Franco Basaglia e mi lasci anche estendere il pensiero a sua moglie e sua compagna di tante battaglie, Franca Ongaro *(Applausi)*, che è stata anche una nostra collega, essendo stata senatrice per due legislature. Nel pochissimo tempo che ho a disposizione voglio dire sostanzialmente due cose per ricordarlo. La prima è che dobbiamo a Franco Basaglia la visione delle persone con malattia psichiatrica come persone e non come malattia. Lui ha teorizzato teorizzato e praticato l'idea che quelle persone avessero la necessità di essere riconosciute in quanto tali, che fosse loro riconosciuta la dignità di persone e che parte della cura fosse partire proprio dal riconoscimento che la persona con una sofferenza psichiatrica non fosse un rifiuto della società, ma qualcuno

la persona un oggetto e non dovesse scalfire in alcun modo la sua umanità e la sua dignità. La seconda cosa che voglio dire è che la conseguenza del riconoscimento della persona con malattia psichiatrica in quanto tale, in quanto essere umano e non in quanto rifiuto, è che non potevano esistere discariche di rifiuti per persone con malattia psichiatrica, perché non erano rifiuti, appunto.

psichiatriche, ma esprimeva una diversità, una marginalità, una non conformità e che in quanto tale veniva considerata degna di essere messa via.

come le carceri o i centri permanenti per il rimpatrio (CPR) dove ci sono persone che non dovrebbero essere lì, esattamente come i malati psichiatrici, o presunti tali, non dovevano essere nei manicomi. Ancora oggi abbiamo delle strutture che servono a risolvere un problema che la società non sa come risolvere diversamente. Se oggi, quindi, ricordiamo Franco Basaglia con sincerità, non possiamo non porci il problema di quelle strutture che oggi ricoprono il ruolo che avevano i manicomi prima dell'arrivo di Franco Basaglia. E dobbiamo interrogarci, dunque, su come gestiamo la marginalità e di quanto nell'altro guardiamo la persona e non il rifiuto umano.

luoghi di guarigione. Erano luoghi, anzi, di uno stigma perenne, la pazzia, che riguardava, almeno per quanto concerne la reclusione, quasi sempre le classi subalterne, i proletari. Già dagli anni Sessanta, però, prima a Gorizia, poi a Trieste, poi un po' alla volta in altri manicomi italiani, cominciava una delle più importanti e profonde rivoluzioni culturali, scientifiche e civili dell'Italia repubblicana: Franco Basaglia, Franca Ongaro - è stata adesso ricordata - l'*equipe* di Gorizia e poi tanti psichiatri, infermieri, assistenti sociali ed anche pazienti ed ex pazienti rovesciarono un paradigma pseudoscientifico che nascondeva un esercizio violento del potere fatto di elettroshock, camicie di forza, letti di contenzione, botte, degrado e che in sostanza riproduceva e spesso produceva quella alienazione che avrebbe dovuto curare. Quella rivoluzione era fatta di scelte semplici ed enormi, come spesso le rivoluzioni vere sanno fare: sostituire la violenza col dialogo e la psicoterapia, aprire porte, abbattere cancelli e sbarre, far uscire i malati nelle città e far entrare la città nei manicomi; feste, socialità, relazioni di cui erano stati arbitrariamente e inutilmente privati, spesso fin da bambini, perché a volte nel manicomio si entrava da piccoli e si usciva da morti, e ancora assemblee di reparto in cui i malati potevano finalmente prendere la parola, esprimere bisogni e diritti. I matti diventavano cittadini malati e cessavano di essere cose, oggetti, numeri. Ma quella liberazione non liberava solo i malati: liberava dal loro ruolo di oppressori anche medici e infermieri e parlava ben oltre le mura degli ospedali psichiatrici dei diritti e delle libertà degli esseri umani e della loro dignità, ricongiungendosi così con le battaglie sociali di quei due formidabili decenni, tra le quali quella contro le classi differenziali e per l'inclusione nelle scuole pubbliche. Semplice e potente, dunque, quella rivoluzione culturale, ma fondata su presupposti insieme scientifici e democratici. La malattia mentale non richiede reclusione, repressione e isolamento, ma al contrario ascolto, socialità, relazione umana e terapeutica, cioè inserimento attivo nel tessuto umano, libertà, umanità e dignità come assi imprescindibili della cura. Franco Basaglia è stato, dunque, un grande scienziato, ma lo è stato perché uomo e cittadino a tutto tondo e non ha mai dimenticato che in una democrazia nessuna scienza e nessuna terapia prescindere dai diritti universali di ogni malato in quanto cittadino e in quanto essere umano. Quella rivoluzione della legge n. 180 del 1978 è stata, però, in larga parte disattesa e tradita. Faremmo un torto a Basaglia se oggi, mentre celebriamo i cento anni della sua nascita, non lo ricordassimo con forza, perché alla critica all'istituzione totale del manicomio essa associava un impegno della Repubblica verso la medicina sociale e del lavoro, verso la medicina territoriale e la prevenzione, una seconda decisiva parte strettamente legata al Servizio sanitario nazionale che, invece, progressivamente, le politiche dei tagli e delle privatizzazioni hanno tradito e allontanato. Per questo noi non ci limitiamo a celebrare Franco Basaglia e, coerentemente con il senso profondo della sua battaglia, abbiamo presentato, a prima firma del senatore Magni, un disegno di legge per una salute mentale di comunità, per garantire a tutte le persone con sintomi di disagio l'effettivo accesso ad un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro esigenze. Per noi ricordare Basaglia significa riaprire la lotta per il diritto universale alla salute, contro ogni mercificazione e contro lo smembramento del Sistema sanitario nazionale. Lo facciamo oggi, con la consapevolezza delle sue parole: la Costituzione vale per tutti, anche per i matti.

Basaglia. Mi occupo dei temi della salute mentale da qualche tempo, e ne ho parlato tante volte in quest'Aula. E se oggi ne parliamo in termini completamente diversi; se parliamo addirittura di avere un'assistenza psicologica nelle scuole; se abbiamo istituito un un *bonus* per il sostegno psicologico dopo i traumi causati a tanti giovani e meno giovani dal COVID o da altre situazioni che vivono quotidianamente; se siamo riusciti a fare questi grandi passi avanti nel nostro Paese, è per le basi che ha posto nel secolo scorso il professor Basaglia, a cui tutti noi dobbiamo rendere onore. *(Applausi)*. È grazie a lui, infatti, che è cambiata completamente la gestione del malato psichiatrico nel nostro Paese, sono cambiati l'approccio e anche il giudizio delle persone nei loro confronti e questo ci ha fatto sicuramente fare dei passi avanti, ma non ci possiamo fermare. Se veramente vogliamo rendergli onore, ora e anche in seguito, dobbiamo portare davvero a compimento i principi della legge n. 180 del 1978, quella che decretò la chiusura dei manicomi, perché in parte ancora oggi è disattesa. Ancora oggi vediamo che i centri di salute mentale, quelli per la gestione territoriale

nascita di Franco Basaglia. Per capire davvero cosa sono stati il suo coraggio e la sua visione, bisogna ascoltare prima di chiunque altro le persone che, in quanto affette da malattia mentale o da disturbo psichico, sono state non solo da lui liberate, ma hanno anche ritrovato la dignità che si deve a ogni donna e a ogni uomo vivente, una nuova dimensione esistenziale. Basaglia ha rivoluzionato la cura della malattia mentale e il mondo della psichiatria così com'era e come l'ha trovato quando è diventato direttore degli ospedali psichiatrici, prima a Gorizia, poi a Colorno e infine a Trieste, dove ha certamente lasciato il segno straordinario di ciò che le istituzioni possono fare mettendo in discussione se stesse in nome di un bene superiore rispetto all'autoconservazione. Questo bene è la dignità, il rispetto della persona, sia essa malata, sana, fragile, forte, povera o ricca. Basaglia ha riconosciuto del manicomio la natura di classe

potesse ritrovare un posto in questa società. C'è voluto un grande coraggio per fare ciò che Basaglia ha fatto, ma ci sono voluti anche un grande, potente cuore e una formidabile intelligenza. Il coraggio di Basaglia, è stato scritto, ha permesso di realizzare l'impossibile, che è diventato possibile; di realizzare non una società senza diversi, ma una società diversa, una società a cittadinanza diffusa. Quale ambizione più grande può avere la politica, se non quella di costruire una società, una comunità, in cui c'è un posto per tutti e per ciascuno di noi? In cui il diritto di cittadinanza è concretamente riconosciuto senza esclusione? Una società che fa della battaglia contro l'esclusione un obiettivo condiviso? Il suo lavoro, straordinario, che ha portato l'Italia davvero ai vertici, all'avanguardia nel mondo, non è certo finito con l'approvazione della legge n. 180 che ha abolito i manicomi. In troppi servizi psichiatrici di diagnosi e cura negli ospedali si adottano, ancora oggi, pratiche di contenzione e forme intollerabili di maltrattamento. Mai come oggi siamo chiamati davvero a dare seguito all'azione e all'intuizione di Basaglia e a fare in modo che la politica metta la salute mentale finalmente al posto necessario e faccia ciò che serve, riprendendo il suo insegnamento. Quella legge fu approvata a larga maggioranza, ma è stata lasciata cadere quasi nel nulla. Io voglio ricordare qui anche lo straordinario lavoro di sua moglie e il lavoro che ancora aspetta e riguarda tutti noi, anche per valorizzare la figura di Basaglia a livello internazionale, a cominciare da quell'archivio importantissimo che è conservato

Ad integrazione e parziale modifica di quanto comunicato in ordine al calendario dei lavori, si informa che giovedì 21 marzo, alle ore 10, al posto delle mozioni avrà luogo un'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I Gruppi parlamentari potranno intervenire per cinque minuti. **Interventi su argomenti

Barbara Balzerani, nota esponente della colonna romana delle Brigate Rosse, condannata all'ergastolo per l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze, Lando Conti, e responsabile, mai pentita e mai dissociata, di azioni come la strage di via Fani e il sequestro Moro. In seguito alla morte di Barbara Balzerani, una docente universitaria, nota a molti anche per le sue frequenti apparizioni televisive,

testualmente: «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia addio alla compagna Luna». Questo *tweet* l'ha scritto Donatella Di Cesare che, oltre che essere nota per le sue apparizioni televisive e anche per partecipare spesso ai corsi di formazione del MoVimento 5 Stelle, è anche docente dell'università La Sapienza di Roma. È vero che nel manifesto del comunismo scritto da Engels e Marx c'è scritto a chiare lettere che i comunisti non disdegnano di manifestare ciò che sono; che dichiarano apertamente quali sono i loro obiettivi e i loro fini, e che questi possono questi essere raggiunti solo con il rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale finora esistente. Però è anche vero che nelle nostre università ci sono tanti docenti e tanti studenti che spesso e volentieri subiscono sanzioni draconiane, certamente eccessive, per aver scritto o fatto molto meno di quello che ha scritto la professoressa Di Cesare. Pochi giorni fa abbiamo letto che Mario Bassani, un importante storico che insegnava alla Statale di Milano, è stato allontanato e che gli è stato sospeso per un mese lo stipendio perché aveva pubblicato un meme offensivo nei confronti della vice presidente Kamala Harris degli Stati Uniti. Qualche mese fa abbiamo letto di studenti della Bocconi di Milano che hanno ricevuto sei mesi di sospensione perché ironizzavano su Instagram rispetto alla

un doppiopesismo negli atenei e nelle università italiane rispetto al comportamento di chi è pagato con i soldi di tutti noi cittadini. Quando cittadini. Quando la Di Cesare dice «la tua rivoluzione è stata anche la mia»; quando dice «le vie diverse non cancellano le idee», vuol dire che Barbara Balzerani per lei non è nemmeno da annoverare tra i cosiddetti compagni che sbagliano - termine caro spesso al giustificazionismo di certa sinistra - ma è semplicemente una militante rivoluzionaria che ha usato, nella lotta armata, un mezzo diverso rispetto a quello che lei evidentemente usa dietro la cattedra. Barbara Balzerani è la stessa che, in occasione dei quarant'anni della strage di via Fani, scriveva su Facebook: «Chi mi ospita oltre confine per i fasti del quarantennale?». Questo è per capire di chi stiamo parlando. Con questo mio intervento, signor Presidente, volevo preannunciare che ho presentato un'interrogazione al ministro Bernini per capire, vedendo che passano i giorni e non c'è notizia di alcun tipo di provvedimento disciplinare nei confronti della professoressa Di Cesare, se l'università La Sapienza di Roma e più in generale gli atenei italiani hanno un doppiopesismo nel giudicare gli atti dei loro docenti. *(Applausi)*. Auspico che ci sia anche da parte del Ministero dell'università un intervento ispettivo per capire cosa per capire cosa vorrà fare l'università La Sapienza di Roma, perché riteniamo che l'apologia degli atti dei terroristi non rientri in quella libertà di espressione alla quale tutti giustamente ci appelliamo e che dobbiamo difendere con ogni mezzo, ma ma che in questo caso è stata ben oltrepassata.

il nome di una donna che è stata colpita da un tumore polmonare non a piccole cellule. È un particolare tipo di tumore, che ha un tipo di farmaco *target* che però ha bisogno, per essere efficace, di un'indagine particolare che si chiama sequenziamento genomico. genomico. È un sequenziamento che consente di comprendere effettivamente la mutazione genetica che ha questo tipo di tumore.

questo fondo non è enorme: di tratta di 5 milioni di euro. Abbiamo parlato di 80 milioni di euro a Cortina, un miliardo per l'intelligenza artificiale. È un fondo di 5 milioni che

non la può fare. Pensateci, pensiamoci. Abbiamo bisogno della vostra sensibilità, della nostra sensibilità. Orsola ha bisogno del sequenziamento genomico. Come Orsola, ci sono 26.000 persone, donne che hanno questo tipo di tumore polmonare non a piccole cellule, a cui non possiamo fornire un'appropriata indagine per poterlo combattere. Manca il fondo.

Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, permette agli